L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

in tempo per consentire ai colleghi di arrivare all'ora prevista per la seduta in Aula, altrimenti tutti i giorni alcuni colleghi, che sono certo stavano lavorando in Commissione, fanno la figura di quelli che arrivano più tardi.

in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», premesso che:

l'articolo 3 di questo decreto-legge al comma 1 prevede risorse per finanziare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità dei giovani solo del Mezzogiorno. I successivi commi disciplinano l'estensione della sperimentazione della cosiddetta nuova carta acquisti del territorio solo nel Mezzogiorno. Mi chiedo come sia possibile che i Ministri di questo Governo riescano a fare un simile provvedimento che discrimina i cittadini del Nord.

Presidente, l'emendamento 3.1 si riferisce ad una diversa ripartizione di alcuni fondi tra varie tipologie di giovani.

dal comma 1 articolo 3, che prevede appunto misure aggiuntive per l'occupazione giovanile. Vengono destinati 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le borse di tirocinio formativo a favore di questi giovani. Ebbene, data la situazione italiana e l'alto tasso di disoccupazione e le difficoltà che incontrano

(ex *social card*) è sperimentata tra le fasce di popolazione che versano in condizioni di maggiore bisogno entro un limite massimo di risorse pari a 50 milioni di euro nei Comuni con più di 250.000 abitanti. I commi dal 2 al 5 dell'articolo 3 dispongono un'estensione della sperimentazione della *social card* nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015,

È un modo per aiutare l'imprenditoria giovanile utilizzando i rifiuti, che in questo momento rappresentano un grande problema per il nostro Paese. All'interno dell'emendamento vengono promosse attività ed azioni per il recupero del patrimonio immobiliare al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore delle nuove imprese. È un modo per recuperare gli immobili italiani ed aiutare la creazione di impresa

alle altre forme di iniziativa legislativa, ma non ai decreti-legge. siamo nel caso di un provvedimento che aveva la relazione tecnica iniziale (quando è stato presentato al ramo del Parlamento che lo ha esaminato per primo) e che passa oggi al Senato. Siccome c'era questo problema di natura regolamentare, la legge n. 196 del 2009 (la legge di contabilità) - questo conferma che era necessario sopperire ad una carenza e normativa sul problema della seconda Camera che esamina il provvedimento - all'articolo 17 ha previsto all'articolo 17 ha previsto che ci sia una relazione tecnica cosiddetta di passaggio, cioè quando si passa dalla prima alla seconda lettura del provvedimento. la legge, in questo caso, di nuovo non ha posto come condizione di procedibilità l'assenza di relazione tecnica: non vi è nel Regolamento, né vi è nella legge. credo che ritenere che non si dovesse procedere all'incardinamento del provvedimento non sia esatto. Abbiamo fatto bene a cominciare ad esaminare il provvedimento, e non vi è una censura né di carattere normativo, né di carattere regolamentare. Questo, signor Presidente, - naturalmente lo dico a conforto della posizione della Presidenza del Senato - non non ci esime dal chiedere, e anche con insistenza, la relazione tecnica, perché riteniamo che ci debba essere il massimo di visibilità della onerosità di tutte le norme, in particolare di quelle che sono state aggiunte durante l'esame presso la prima Camera. Lo stiamo facendo e la otterremo, naturalmente, in particolare prima dell'esame degli emendamenti (ovviamente è così). In questo senso, ci impegniamo con tutto il Senato, con i colleghi e ancor prima di tutto con lei, signor Presidente, perché le Commissioni riunite 1a e 5a abbiano la relazione tecnica di passaggio per poter verificare le eventuali onerosità e sottoporle a lei anche nella lettura prima dell'Aula. Quindi, nessuna violazione è stata in alcun modo commessa; ma siamo impegnati, sul piano della sostanza, a far sì che la Presidenza del Senato e il Senato tutto abbiano piena cognizione dell'intero provvedimento e dei suoi caratteri di onerosità.

il presidente Azzollini per le precisazioni e mi scuso, perché noi siamo appena arrivati e lei sicuramente è più esperto di noi. Volevo soltanto porre un altro quesito. Da quello che avevo capito io, la relazione tecnica, per quanto riguarda il passaggio tra i due rami del Parlamento,

aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento». Le condizioni di procedibilità non possono che essere espresse e puntuali, perché tipiche: non c'è la condizione di improcedibilità e, quindi, io sono

a porre in essere ogni attività per l'inserimento del reddito minimo garantito,

il testo provvede a dare risposta alle condizioni di povertà assoluta in cui si trova la popolazione del Mezzogiorno che, secondo i dati ISTAT, ha un'incidenza più che doppia rispetto al resto del Paese.

sia come singolo, sia nelle formazioni sociali...». All'articolo 3 è previsto che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge...» e che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli» - e la la povertà sicuramente è un ostacolo - «di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...».

Quindi, chiaramente, nel momento in cui vi è una situazione di ristagno economico particolarmente rilevante come quella che è stata messa in evidenza dall'ISTAT, è compito della Repubblica rimuovere... PRESIDENTE. La invito Grazie

*(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei ringraziare la collega Nugnes perché ha voluto leggere la Costituzione. È evidente che la Costituzione per la collega vale solo per il Mezzogiorno, perché lei ha letto esattamente quello che c'è scritto, e le volevo ricordare che quello che c'è scritto vale per tutto il Paese, come ha letto lei.

ogni volta che si affronta la questione legata al lavoro, si tende sempre ad individuare il Mezzogiorno come area da sostenere perché individuata come area in difficoltà, quando sappiamo bene che è un'area che ha delle risorse enormi e potrebbe essere assolutamente parificata al Settentrione, quindi a tutta l'Italia. Pertanto, dal mio punto di vista, è possibile sostenere l'emendamento 3.200 della Lega, Lega, con la soppressione nell'articolo, della specificità del Mezzogiorno, lasciando quindi che tutto l'articolato del decreto-legge intervenga in termini generali su tutto su tutto lo Stato, senza differenziazioni specifiche. Sull'emendamento 3.201 invece no, ovviamente, in quanto esso sostituisce il Mezzogiorno con la Macroregione del Nord, quindi andrebbe ad invertire qualcosa per

*(PdL)*. Signor Presidente, avevo ricordato già nella seduta di ieri per la verità che il voto in dissenso non può essere accompagnato da motivazione. Il senatore che dissenta rispetto al voto del proprio Gruppo si deve limitare ad esprimere il suo dissenso, la contrarietà, e non impegnare del tempo in quest'Aula per spiegare delle motivazioni che per il Regolamento non sono dovute. devo assolutamente rispondere, perché l'articolo 109,

«è riconosciuta ai senatori che intendono dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso». Quello cui si riferisce il senatore Falanga è la dichiarazione di voto uguale a quella del Gruppo, che può essere fatta, espressamente, dicendo sì o no; uguale facoltà si intende che prima di ogni votazione si può svolgere una dichiarazione di voto a nome del Gruppo per non più di dieci minuti.

vorrei dichiarare il mio voto contrario all'emendamento 3.203 a prima firma Munerato, perché ancora una volta, seppur di poco, si vanno a tagliare dei fondi per le infrastrutture e la valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno.

Signor Presidente, l'ostruzionismo è una pratica nobilissima, ma non può scendere nella farsa, e lei deve garantire l'Aula che non scendiamo

Senatore Santangelo, la sua lettura contraddice quello che vuole sostenere, perché vale nelle votazioni per alzata di mano; quando lei chiede la votazione con sistema elettronico, il discorso può non valere. Quindi scelga lei.

vorrei capire se, dal punto di vista regolamentare, la richiesta di voto elettronico può essere formalizzata senza alcuna richiesta verbale

Vorrei capire se per richiedere il voto elettronico basti un cenno che chiunque dei senatori può fare al Presidente in modo da snellire questa prassi antipatica, non soltanto per me.

perché voi avete dovuto rivedere il testo con una relazione tecnica aggiuntiva e avete votato contro a quanto io chiedevo nell'emendamento e che poi vi ha portato a

Gli emendamenti intendono precisare che tale nuova struttura, che opera in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, non deve comportare oneri aggiuntivi per lo Stato, ma soltanto rimborsi di eventuali e documentate spese di missioni, visto che sarà coordinata dal segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale e sarà composta dal presidente dell'ISFOL, dal presidente di Italia Lavoro SpA, dal direttore generale dell'INPS e dai dirigenti generali dello stesso Ministero del lavoro; naturalmente trattasi di di dirigenti già ben remunerati. I nostri emendamenti prevedono, conseguentemente, la soppressione del comma 4 che pone la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della neostruttura: 40.000 euro per il 2013 e 100.000 euro per il 2014 e 2015 a carico del Fondo sociale per l'occupazione. In un periodo di forte crisi economica, con la necessità di reperire risorse per gli ammortizzatori in deroga e soprattutto per salvaguardare gli esodati, esodati, con l'obiettivo di risparmiare e contenere i costi della spesa pubblica è impensabile prevedere nuove strutture composte da burocrati dello Stato con importanti oneri e costi ulteriori.

il caso di Italia Lavoro SpA e dell'ISFOL è interessante in quanto si tratta di due strutture dedicate al servizio del mercato del lavoro, sulla cui efficienza e congruenza dei costi in termini di risultati e di efficacia degli interventi sono stati sollevati numerosi dubbi. Noi chiediamo che questa sia l'occasione per mettere in modo rigoroso sotto controllo tale incongruenza. L'emendamento 5.202 mira a questo. Confido che tale intendimento sia condiviso dai relatori e dal Governo.

riorganizzazione dei servizi per l'impiego

dei quali non si conoscono efficacia ed efficienza, non si capisce quindi per quale motivo questi servizi debbano essere effettuati, ancor prima delle valutazione degli stessi, proprio da quelle società.

L'ordine del giorno G5.101, presentato dalla senatrice Catalfo,

Dichiaro aperta la votazione.

che rispecchia una considerazione su cui tutti sono concordi, e cioè il nostro sistema della formazione professionale finanziata con denaro pubblico soffre di un grave difetto: la mancata rilevazione sistematica del tasso di coerenza tra formazione impartita e risultati occupazionali conseguiti. Tale rilevazione, relativamente facile sul piano operativo e poco costosa, può essere realizzata con estrema facilità utilizzando il personale di cui disponiamo. L'unico motivo per non rilevare questo dato è la volontà di non evidenziare situazioni di gravissima inefficienza e inefficacia

realizzare valutazioni dell'efficacia e dell'efficienza che richiedono - lo ripeto ancora una volta - strumenti statistici approfonditi e sofisticati che, a loro volta, comportano un finanziamento consistente. Ciò che si può trarre da questo emendamento è un ordine del giorno che inviti il Governo ad intensificare la propria attività

relativo alle modalità di rilevazione dei dati concernenti l'attività formativa che, com'è noto, è in capo alle Regioni. viene sviluppata attraverso un contributo significativo delle dotazioni finanziarie di provenienza comunitaria

dello sviluppo da realizzare, quindi la valutazione dei fabbisogni formativi non è possibile perché non sappiamo cosa dobbiamo produrre, come e dove lo dobbiamo produrre. Aver lasciato tutto in mano al mercato significa non poter fare programmazione dal punto di vista della formazione, di quella professionale, di quella alta che serve a dare innovazione al nostro Paese. Per questo voteremo

un'analisi approfondita di questo settore, dei risultati che realizza, ma soprattutto delle coerenze che deve realizzare rispetto ad un'idea di sviluppo che purtroppo ancora manca a questo Paese.

che non siamo in grado, se non aggiungendo risorse al funzionamento di istituzioni che in parte sono dedicate a questa missione, di svolgere un'attività preliminare

Signor Presidente, non posso che ripetere quello che ho detto. Un emendamento di questo tipo prevede un'attività di valutazione per tutti i corsi di formazione professionale che assolutamente non può essere fatta con pochi dipendenti

con gli strumenti adeguati, penso che, una volta demandata al Ministero del lavoro e alle sue agenzie, questa potrebbe essere in tutti i Paesi del Centro e del Nord Europa ogni centro di formazione professionale, ogni facoltà universitaria pubblica il dato relativo agli sbocchi occupazionali di chi ha completato il corso o ha conseguito il diploma *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ciò consente a chi compie le proprie scelte di formazione di sapere qual è la probabilità, frequentando quel corso, di ottenere un'occupazione coerente con il suo contenuto. Questo, in realtà, potrebbe essere ottenuto semplicemente vincolando ogni struttura di formazione ad intervistare a tre mesi o a sei mesi dalla fine del corso il proprio diplomato. Abbiamo centinaia ma anche migliaia di collocatori, di addetti ai centri per l'impiego. Se non cominciamo a svolgere quest'attività non arriveremo mai a svolgerla in modo compiuto. Il Sottosegretario ritiene che questo progetto sia troppo ambizioso, ma se non cominciamo a proporci qualcosa di ambizioso nel mercato del lavoro, avremo sempre un mercato del lavoro in coda rispetto a tutte le graduatorie di efficienza sul piano europeo, ma ormai anche su quello mondiale. sociali*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 5.203 per trovare una formulazione che possa soddisfare il Governo e il Parlamento.

le esperienze, purtroppo ancora molto rare, di alternanza tra scuola e lavoro sin dal primo anno delle scuole superiori, e quindi anche dal quattordicesimo anno di età. Non si tratta di rapporto Non si tratta di rapporto di lavoro, ma si tratta di esperienza in ambito lavorativo che concorre all'educazione della persona appunto - il lavoro deve essere ritenuto parte del processo formativo. Non si comprende il motivo per cui nel primo anno delle scuole superiori non possa già avviarsi ciò che purtroppo viene praticato ancora in misura molto contenuta, cioè l'interazione tra l'apprendimento teorico e l'esperienza pratica in contesto lavorativo.

dei giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Ciò è doveroso in un decreto che si propone di favorire l'occupazione, specie quella giovanile. Pertanto, invito ancora una volta il Governo ed anche i senatori che hanno firmato l'ordine del giorno G2.100 a valutare con favore

qualche migliaio di persone da anni in balìa dell'insicurezza e dell'incertezza e nei confronti della quali è stata dichiarata da più parti l'opportunità di una stabilizzazione, non solo ai fini di una migliore funzionalità degli istituti, ma anche ai fini di un risparmio economico vero e proprio. L'altra volta con il Governo vi fu un *qui pro quo*

attraverso un'esternalizzazione del lavoro, vengano finalmente inglobati nell'organizzazione scolastica. Sono appunto servizi che normalmente la scuola

Presidente, trovo che non approvare l'emendamento 7.13 sia un atto grave ed antidemocratico. Ora, io non pretendo che i lavoratori debbano essere ascoltati e capiti come meriterebbero, mi rendo conto, purtroppo, che gran parte di questa politica non ha voglia di farlo, ma che addirittura si voglia negare la possibilità ai lavoratori di votare sulle proprie condizioni tramite *referendum* e per giunta a costo zero è da considerarsi, a mio avviso, per la serie: come continuare ad offendere l'intelligenza dei lavoratori.

massimo di 36 mesi con lo stesso datore di lavoro, nell'arco di tutta la vita lavorativa. Ci sono alcuni lavoratori che purtroppo, una volta cessati i 36 mesi con un'azienda, non riescono a trovare altri lavori

l'emendamento 7.203. Il comma 1 dell'articolo 7 contiene modifiche alla disciplina del contratto a termine. Il presente emendamento che sopprime il numero 1), della lettera *d)* di tale comma è finalizzato a prevedere la possibilità che i contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori iscritti alle liste di mobilità possano essere privi di causale e quindi derogare al principio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sul punto, la giurisprudenza si è già espressa affermando che la fattispecie in questione deve essere ricondotta alla disciplina generale stabilita dal suddetto decreto legislativo, con la conseguenza che in difetto del collegamento causale anche il termine apposto ad un contratto stipulato con un lavoratore iscritto

l'emendamento 7.204 mira a consentire l'utilizzazione del contratto di lavoro intermittente nel settore del turismo, cui le esigenze che possono dar luogo a una legittima e utile attivazione di tale contratto sono abbastanza evidenti. Chiediamo dunque che il Governo e i relatori

all'agevole continuazione di collaborazioni a progetto, ove il programma di ricerca sulla stessa materia o per materie affini abbia a proseguire. la nostra proposta relativa ad un uso più agevole dei buoni prepagati - o *voucher* - per la regolarizzazione di spezzoni lavorativi, in modo particolare in agricoltura. Le disposizioni della legge Fornero hanno irrigidito l'impiego dei buoni prepagati che, purtroppo, è ancora molto limitato. Non siamo, cioè, in presenza di una possibile patologia da inflazione dello strumento, che è in realtà impiegato soltanto in una parte del Paese: sotto la "linea gotica" sfuma, fino a sparire completamente. Dovremmo preoccuparci di quegli ambiti lavorativi, soprattutto nel settore agricolo, ove non vengono impiegati i buoni prepagati e non delle aree nelle quali lodevolmente hanno consentito

e ricordare che nell'ambito dell'industria discografica tutti i cantanti sono associati in partecipazione e, d'altronde, questa si rivela essere la modalità più coerente con cui regolare il rapporto di lavoro tra l'artista e la casa discografica. Peccato che, non so se in omaggio a qualche rito esoterico, la legge Fornero abbia introdotto il limite di tre per le cosiddette associazioni in partecipazione, a prescindere dalla loro caratteristica genuina o meno. Nella mia cultura il tre non ha nessun significato; forse a Torino la cosa è diversa. Chiedo davvero di superare questo limite, quanto meno nell'industria discografica. Sarebbe ridicolo se oggi un ispettore del lavoro entrasse in una di queste aziende e trasformasse *ope legis* Vasco Rossi in un lavoratore subordinato. Ma tant'è: questo accade

solo l'emendamento 7.211. L'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, modifica il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio. Il corrispettivo, infatti, non è più esclusivamente rimesso alla libera negoziazione delle parti in relazione al valore di mercato della prestazione, ma è legato ad un parametro orario di durata della prestazione stessa. In particolare, è previsto che una prestazione accessoria di durata di un'ora debba essere remunerata almeno con un *voucher*, attualmente del valore di dieci euro. Questa previsione contrasta con i principi generali del nostro ordinamento secondo i quali il compenso per lo svolgimento di un'attività di lavoro non dipendente, come il lavoro accessorio, è legato al valore dell'opera o del servizio che viene eseguito e non alla durata della prestazione. Inoltre, il valore nominale di un buono pari a dieci euro appare eccessivo per un'ora di lavoro rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva per analoghe prestazioni rese dai lavoratori dipendenti e rischia di porre fuori mercato il lavoro accessorio in agricoltura.

superando l'orientamento dei precedenti interventi legislativi che hanno pensato di risolvere la crisi occupazionale ed economica aumentando la flessibilità in uscita ed erodendo le garanzie dei lavoratori. Con questo emendamento proponiamo di ripristinare il testo originario dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in vigore prima dello stravolgimento della legge Fornero, la n. 92 Riteniamo che la nozione giuridica secondo la quale nessuno può essere licenziato senza giusta causa o giustificato motivo debba essere al più presto pienamente ripristinata. La reintegrazione nel posto... *(Il microfono si

ma siamo sottoposti ad uno *stress* da «normificio» che non ci consente neppure di ragionare su quello che stiamo votando. Siamo stati investiti del decreto «del fare» ieri notte e dobbiamo presentare gli emendamenti entro le ore 20. Contemporaneamente siamo in Aula a votare un altro provvedimento con ritmi di questa natura.

per cui quando si tratta di contrattazione aziendale, territoriale, nazionale che riguarda i diritti dei lavoratori si fa il *referendum*, oppure ogni *referendum* che si fa è privo di ogni valore a giustificazione di una politica. In questi anni - e la vicenda FIAT ne è stata una testimone una testimone - il *referendum*, utilizzato, anche strumentalmente, per escludere i lavoratori in violazione di norme costituzionali,

È un atto di democrazia e noi non dobbiamo dimenticare tutta la democrazia e tutta la cultura democratica di cui siamo espressione! ogni modifica che proponiamo non è accolta. E ogni attenzione che proponiamo non è accolta!

questo emendamento riguarda la possibilità di utilizzare il lavoro intermittente nel settore del turismo. Mi risulta che su questo emendamento ci sia un larghissimo consenso, non solo

Ricordo che se non ci fosse il lavoro intermittente non ci sarebbe lavoro in questi comparti, che tra l'altro - lo ricordo - non hanno magazzino:

In questo senso,

in esame si riferisce soprattutto ai casi delle cooperative sociali che utilizzano detenuti all'interno delle carceri: quando finisce la detenzione,

lei lo ha dichiarato improcedibile, però non mi risulta, perché è una questione totalmente burocratica che il Ministero si è assunto

sulla dichiarazione di preclusione di un emendamento. Io non sono il presentatore dell'emendamento, io sono un senatore come tanti altri presenti in quest'Aula.

intendo è l'opportunità di avere chiarezza su quello che stiamo votando, su ciò che viene precluso e sui motivi. Sinceramente, non avendo conoscenza diretta dell'emendamento del collega Puglia e andandolo a leggere, noto che l'emendamento 7.216 è completamente diverso rispetto al precedente: e vedere che si va avanti senza una motivazione credo che sia mortificante per tutti. Oggi capita a noi, ma quanti emendamenti sono stati preclusi o dichiarati improcedibili senza uno straccio di motivazione, almeno minima? Questo sto chiedendo, e lo faccio a nome di tutti,

l'emendamento 8.0.1 tende a sopprimere la società Italia Lavoro Spa

parlano, che gli stessi servizi per l'impiego siano efficaci ed efficienti. Al fine di valutare la congruenza di tutto quello ad oggi fatto

del decreto-legge, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 9.213, 9.53, 9.0.1, 10.200 e 10.202, nonché gli ordini del giorno G9.108 e G9.109, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

normale e cortese.

sottolineare due obiettivi molto cari al Movimento 5 Stelle. Il primo obiettivo è eliminare i conflitti di interesse, il secondo, ancor più importante (penso per tutti), avvantaggiare e dare sostegno alle piccole imprese. si propone di dilazionare gli aumenti delle sanzioni

È comprensibile, in questo momento di crisi delle aziende, cosa può rappresentare un aumento di quasi il 10 per cento delle sanzioni per le aziende.

quello di diploma professionale. Il presente emendamento è finalizzato alla soppressione della disposizione che consente la trasformazione di questo contratto di apprendistato per la qualifica e diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante. Questo non è assolutamente corretto. Il periodo scolastico attiene alla fase di formazione scolastica - vi invito un attimo

intendo illustrare l'emendamento 9.93, che riguarda il telelavoro, in Italia ben poco praticato. poco praticato. Lo Statuto dei lavoratori nel 1970 - e pensate alle tecnologie del tempo - ha disposto il divieto di qualsiasi tecnologia che comporti controllo a distanza. È una norma per molti aspetti obsoleta, evidentemente; è sufficiente avere un'auto aziendale con il satellitare incorporato per essere in una condizione

Qui si dice che, almeno per il 50 per cento, queste tecnologie di controllo a distanza devono poter essere limitate in modo da rendere compatibile il telelavoro,

mettere in discussione l'articolo 4 di una legge del 1970, che comunemente chiamiamo Statuto dei lavoratori. [DI

preventivamente dell'improcedibilità. Siccome ho provveduto al ritiro, che è stato naturalmente ininfluente, vorrei capire come regolarmi per gli articoli a seguire.

Signor Presidente, con l'emendamento 9.94 noi chiediamo di prevedere per le cooperative della piccola pesca una differenzazione rispetto a quanto proposto dall'articolo 7, nella legge n. 31 del 2008, poiché trattasi di una fattispecie molto particolare. Immaginare di sottoporre le cooperative della piccola pesca allo stesso schema della contrattazione collettiva nazionale

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9 tende a dire che, laddove il contratto collettivo abbia escluso la responsabilità solidale tra appaltatore e committente, questa esclusione vale soltanto per la retribuzione ma non per la contribuzione previdenziale relativa a questa retribuzione. Questo significa il committente verrebbe esonerato dalla solidarietà passiva con l'appaltatore soltanto per il debito retributivo ma non per il debito contributivo. Questa è palesemente un'assurdità, perché laddove vi sia esenzione di responsabilità per il debito retributivo, logica vuole che l'esenzione valga anche per il debito contributivo.

Il blocco della sanzione fino al 2015 è comunque una sorta di deterrente per non aumentare il peso della vessazione.

da 102.000 tonnellate, ha sfiorato la collisione con Riva dei Sette Martiri, stringendo verso la banchina un vaporetto pubblico. Già il 7 maggio, al porto di Genova, abbiamo visto la nave "Jolly Nero" distruggere la torre di controllo, uccidendo 9 persone. Aveva una stazza di 40.000 tonnellate, meno della metà della "Carnival Sunshine", che avrebbe potuto schiacciare il vaporetto come un guscio di noce, con tutte le persone a bordo. «Quel vaporetto non doveva trovarsi lì» è stato commentato, ma è la "Carnival Sunshine" che non doveva trovarsi là. Queste navi stazionano per lunghi periodi con ciminiere fumanti a ridosso del centro storico; salpano con migliaia di tonnellate di gasolio nei obbligano a collocare le paratie del Mose a doppia profondità, aumentando enormemente i costi e il flusso di marea che erode i fondali della laguna, ma soprattutto mettono a repentaglio un'intera città. Dopo la tragedia della "Costa Concordia" all'isola del Giglio, i ministri Passera e Clini emanarono un decreto per vietare i transiti in zone sensibili. Per Venezia istituirono un divieto, che però fu subordinato e posticipato alla realizzazione di alternative. Ebbene, ad un anno e mezzo dal decreto non abbiamo ancora un progetto chiaro. Il 12 giugno scorso ho depositato in merito l'interrogazione con carattere di urgenza 3-00127 e mentre attendo risposta accade questo allarmante episodio.

Ben venga se questo favorirà il venire alla luce degli scandali delle opere pubbliche in Veneto e Laguna di Venezia. Abbiamo visto l'arresto di Piergiorgio Baita, presidente di Mantovani Spa, e Claudia Minutino, segretaria del governatore Galan. Ora quelli di Federico Sutto (ex segretario di Gianni De Michelis), Pio Savioli, e soprattutto Giovanni Mazzacurati, consiglieri ed ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico proprio per il Mose,

possibilità alternative o quanto meno il progetto meno oneroso e più collaudato. E magari comprenderemo perché, per risolvere il problema della grandi navi, la maggior parte dei progetti continua a mantenere le banchine di attracco in laguna, scavando enormi canali alternativi, costruendo nuove isole, con costi e impatti ambientali enormi, talora senza risolvere i problemi della navigazione interna. Noi vogliamo soluzioni e vederci chiaro su queste Presidente, colleghi, l'intero Gruppo Movimento 5 Stelle, dicendo no ad ogni violenza da ogni parte provenga, esprime solidarietà agli attivisti No TAV sottoposti a perquisizione delle loro abitazioni con l'infondata, esagerata e irragionevole accusa di attività eversiva collegata al terrorismo. Questa è un'accusa che non sta in piedi e di certo, se non fosse infondata, si esplicherebbe con arresti e provvedimenti detentivi immediati, non con perquisizioni e sequestri di semplici *personal computer* e telefonini. Non siamo più di fronte allo Stato che difende se stesso, ma ad un utilizzo strumentale degli apparati statali, impiegati ad uso e consumo di pochi. questi pochi sappiamo bene chi sono: una ristretta oligarchia infiltratasi nel nostro Stato che difende, con ogni mezzo e strumento, l'interesse economico che sta dietro al TAV. Anche qui viene in mente il caso Shalabayeva, siamo nella stessa situazione: le nostre istituzioni schiave di altre forze, altre potenze, altri interessi. Saccheggiano le nostre risorse non per la costruzione di un'opera con finalità il bene del cittadino, ma per scomporre un enorme flusso di denaro in rivoli più piccoli che abbeverano nicchie di potere e malaffare. Si pensi ai 150.000 euro spesi in dieci mesi per la fornitura dell'acqua utilizzata dai bagni posizionati al cantiere o ai 175.000 euro spesi, sempre in dieci mesi, per la pulizia di 18 moduli *container* o, infine, all'affidamento dei lavori (per importi superiori a 150.000 euro) ad aziende prive dell'attestazione SOA, come invece è previsto dalla legge italiana. Si pensi all'articolo 10 dell'Accordo italo-francese del gennaio 2012 (Diritto applicabile), che prevede la cessione di sovranità da parte dello Stato italiano in quanto tutti gli aspetti salienti della realizzazione dell'opera saranno regolati dal diritto francese. In tal modo si potranno bypassare le regole previste dalla legislazione italiana antimafia (non presente nel diritto francese), le certificazioni obbligatorie per la partecipazione agli appalti e così alla faccia dei protocolli antimafia sottoscritti in pompa magna dalle parti interessate. Se mai arriverà in quest'Aula il disegno di legge di ratifica dell'accordo bilaterale del gennaio 2012 e voi colleghi lo approverete, sarete complici di una di queste grandi truffe perpetrate...

Prego. di morte che accade nel nostro mar Mediterraneo, presso le nostre coste. In particolare, faccio riferimento a ciò che è accaduto nei giorni scorsi in Sicilia, dove l'ennesimo sbarco di uomini, donne e piccoli che scappano da una situazione di miseria o da persecuzione politica sembra quasi non interrogarci più; sembra quasi ci sono stati dei morti in questo mar Mediterraneo, che è stato culla di incontro, d'integrazione di culture diverse che nei millenni hanno lasciato tracce incredibilmente belle

dell'Unione europea si possa parlare di tutto questo, perché è un fenomeno che ci riguarda ogni giorno. Spesso i morti sono dimenticati come si fossero morti di serie B. È un problema drammatico, come se le nostre coscienze fossero quasi prese prese da un'anestesia incredibile, come se tutto il resto ce lo fossimo scordato, come se un Paese di grande civiltà come il nostro avesse rimosso tutto questo. Credo che in questo prossimo semestre il nostro Presidente e il Governo che sosteniamo debbano porre all'attenzione dell'Europa un maggiore un maggiore interesse di tutti, perché non è un problema solo delle nostre coste e del nostro Paese, ma è un problema europeo, affinché si metta al centro l'accoglienza dell'altro. Approfitto di questa occasione per pregarla, signor Presidente,

È un ritardo difficile da giustificare, perché in questo caso non si completa l'attività e il lavoro delle due Aule di Camera e Senato. Essendo in previsione di una convocazione del Consiglio di Presidenza e conoscendo la sua sensibilità, le chiedo, signor Presidente, di farsi portatore di questo indirizzo all'interno del Consiglio di Presidenza medesimo e, se fosse ritenuto opportuno, di informare chi le parla e l'Assemblea delle ragioni di questo ritardo e di come si intende provvedere.

Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, mi preme richiamare l'attenzione di quest'Assemblea sull'ennesimo scempio che si sta perpetrando ai danni del territorio siciliano e della popolazione di tutta la Regione Sicilia per mano della Marina militare statunitense e con il supino consenso del Governatore della Regione Sicilia e di questo attuale Governo. L'ormai nota revoca della revoca emanata dal presidente Crocetta senza neanche consultare l'Assemblea regionale siciliana elimina qualsiasi impedimento al completamento dell'impianto di comunicazioni satellitari della Marina militare statunitense, conosciuto da tutti come MUOS (*Mobile user objective system*). L'impianto, che sorge a ridosso dell'abitato di Niscemi in una zona densamente popolata e per di più all'interno di un'area naturale protetta (la Riserva regionale della sughereta), unica rimasta in tutta l'area del Mediterraneo, fa parte di un sistema di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza a scopo militare. L'installazione militare statunitense insiste su un territorio già duramente provato dalla presenza ormai più che ventennale di un impianto di comunicazioni militare statunitense formato da ben 41 antenne e dalle esalazioni prodotte in oltre cinquant'anni di attività dal polo petrolchimico di Gela. Come spesso accade in questi casi, la popolazione locale è stata tenuta per lungo tempo all'oscuro del progetto e non è stata fornita alcuna informazione sui possibili rischi sanitari legati alle emissioni elettromagnetiche di tali antenne. Soltanto la pressione dei comitati di cittadini preoccupati per la propria salute ha spinto gli amministratori locali a rivolgersi a tecnici esperti per ottenere un parere scientifico sulla pericolosità delle emissioni dell'impianto. Le conclusioni della relazione prodotta dai tecnici del Politecnico di

Non sono d'accordo con queste conclusioni, invece, gli esperti dell'Istituto superiore di sanità nella cui relazione, a volte lacunosa e superficiale, vengono riportati valori delle emissioni elettromagnetiche quasi sempre al di sotto della soglia massima consentita. Movimento 5 Stelle esprime solidarietà nei confronti dei cittadini niscemesi e siciliani che con ogni mezzo si stanno battendo per impedire la realizzazione di questo impianto e si schiera accanto ai colleghi portavoce dell'Assemblea regionale siciliana

ricordare che, proprio mentre era in corso la seduta, si sono svolti a Ravenna i funerali del cardinale Ersilio Tonini, arcivescovo emerito di Ravenna, giornalista, scrittore, filosofo, uomo colto e uomo di dialogo.

apprezzare la sua umiltà, la sua determinazione e la sua disponibilità, sempre, al confronto, che lo hanno reso una persona importante, un punto di riferimento per tanti cittadini italiani, credenti e non credenti, che hanno visto in lui una persona seria che non soltanto proponeva le sue idee, ma che anche testimoniava coerentemente i suoi valori. Quest'oggi è stato ricordato come «pacificatore provocante e riconciliatore coraggioso». Credo che noi tutti in quest'Aula, credenti e non credenti, possiamo guardare all'insegnamento di pace e insieme di coraggio che il cardinale Tonini ci ha trasmesso nella sua lunga vita e nella sua grande e determinata esperienza al servizio del bene comune. ringrazio, senatore Olivero, per questo atto opportuno e doveroso. La Presidenza si associa nel ricordare una personalità così importante nella vita pubblica italiana, per i credenti e per i non credenti, come il cardinale

vorrei esprimere la massima solidarietà del nostro Gruppo parlamentare e la più sincera vicinanza ai consiglieri comunali Novi e Fuggetta del Movimento 5 Stelle di Monza che, in occasione del consiglio comunale di ieri sera, hanno ricevuto una lettera anonima dal contenuto fortemente minatorio. Seconda la lettera, il consigliere Novi è ritenuto colpevole di attaccare la caparbietà di un ente pubblico a difendere un interesse privato, che è quello di chi gestisce l'autodromo nazionale di Monza. Nella lettera consegnata in Comune, un anonimo praticante dello sport automobilistico e sedicente importante imprenditore minaccia: «Attento a come ti muovi. Sappiamo dove abiti e possiamo spaccarti le gambe quando vogliamo». Anche l'altro consigliere è stato avvisato in conclusione della lettera: «Sei amante della cultura araba, popolo da sterminare. Sarai tenuto nel mirino e poi colpiremo». Questo episodio in Brianza mostra che le denunce puntuali dei cittadini sullo scempio della cosa pubblica, dei territori così apparentemente sgombri da affari collusi con il malaffare, stanno producendo effetti finalmente positivi e la strada è quella giusta. Rispondiamo alle intimidazioni con la partecipazione e la mobilitazione affermando quei valori e principi di trasparenza e legalità che mai nessuna casta imbavaglierà. In conclusione, chiedo la solidarietà ai consiglieri comunali Novi e Fuggetta da parte di quest'Aula.

una valutazione politica di indifferibilità, che venga calendarizzato nei tempi più brevi il disegno di legge n. 134 del collega Malan, trattato congiuntamente al disegno di legge n. 642 del collega Casson, in materia di geografia giudiziaria. Evidenzio che la Commissione di merito, la Commissione giustizia, ha approvato un testo dando il mandato al relatore a riferire in Assemblea. La necessità, Presidente, che anche lei ponga i suoi buoni uffici per la salvaguardia dell'autonomia del Parlamento dipende dal fatto che, calendarizzando questo disegno di legge, eviteremmo che la vigenza prevista per il 13 settembre determini una serie di patologie nell'amministrazione della giustizia derivante dall'inopinata